interessa moltissimo la nostra Commissione e l'intero Senato. Da questo ne deriva una forte volontà politica, che intendiamo mettere in atto affinché l'Italia sia attore con

Per quanto riguarda l'Italia, ministro Galletti, si ritiene indispensabile assicurare già fin da ora certezza normativa alle imprese, in particolare sull'*end of waste*, espressione

proponendo il tema dell'economia circolare come centrale, come fattore culturale preventivo, compresa anche la definizione dell'impiantistica necessaria ad attuare questa politica e a valutare il corretto smaltimento del riciclo. come siamo messi da questo punto di vista e se sia in essere un'attività del Ministero affinché si possa lavorare ad una legge quadro nazionale, che ci veda attori complessivi nel settore dei rifiuti.

raggiunto e realizzato. Ovviamente le variabili in campo sono diverse sia per quanto riguarda il valore dei prodotti e dei materiali sia per quel che concerne il ciclo dei rifiuti, di difficile realizzazione, specie nelle grandi città. Sappiamo che, per assurdo, i Comuni cosiddetti ricicloni sono, quasi sempre, quelli che hanno il maggiore prelievo fiscale della TARI sui propri cittadini. La mancanza di un mercato efficiente delle materie prime secondarie è probabilmente il primo freno alla economia circolare. Sappiamo che alla economia circolare sono dedicati, in sede europea, vari atti e strumenti, dal progetto Orizzonte 2020, al Fondo europeo per gli investimenti strategici, alle politiche di coesione, ai fondi regionali. Quindi prevale sinora una visione che sembra puntare innanzitutto sul rifiuto industriale o dei siti produttivi, un ambito, però, ove il recupero di materia prima secondaria costituisce purtroppo un costo improprio per le aziende. Abbiamo l'impressione che manchi una strategia a partire dal basso, cioè dal momento della raccolta della mole principale di materia prima da inserire nell'economia circolare,

Comuni virtuosi dal punto di vista del riciclo. Vorrei inoltre sapere quali sono le iniziative per non oberare di ulteriori oneri le imprese, agevolandone, ove possibile, una pratica di riutilizzo di materie prime secondarie attraverso l'utilizzo delle agevolazioni fiscali. la domanda è unica: come si pone l'Italia rispetto alla valutazione del nuovo pacchetto dell'economia circolare, anche con la dovuta attenzione agli impegni di COP21, visto che la valutazione che sta emergendo in Commissione dal

una deroga pericolosa per i Paesi dell'Est, che potranno avere una proroga di ulteriori cinque anni, quando il 65-70 per cento è un obiettivo che molti Paesi europei hanno già attualmente raggiunto.

c'era l'idea di eliminare il recupero energetico come valutazione di recupero di materia. Stiamo andando verso una direzione diversa da quella degli obiettivi anche per lo spreco di cibo;

Signor Presidente, il 2 dicembre dello scorso anno la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare. Anche l'Italia ha condiviso tale scelta strategica in favore dell'economia circolare, nell'ottica di uno sviluppo che sia sostenibile e, in prospettiva, a rifiuto zero e decarbonizzato. Si tratta di una scelta che, tra l'altro, è condivisa a livello globale dopo l'intesa sul clima siglata nel COP21 di Parigi nel dicembre scorso. La fiscalità energetica ed ambientale, infatti, può rappresentare una leva di sviluppo del lavoro e della competitività del sistema Europa, avviando la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio, elevato risparmio energetico, ridotto consumo di acqua e alta riciclabilità. Penso, ad esempio, alla possibilità di prevedere l'introduzione di benefici fiscali quali aiuto all'investimento in tecnologie a basso impatto ambientale anche nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati, ciò anche al fine di attivare

potrebbe essere interessante riservare una specifica progettualità al trattamento dei sottoprodotti industriali derivati, ad esempio, dalla lavorazione di oli vegetali, di grassi animali e di produzione dei biocombustibili, individuati da norme tecniche. L'eventuale inserimento di questi nel ciclo virtuoso di riduzione dell'impatto ambientale conseguirebbe altresì il valore aggiunto proprio di favorire quei processi di economia circolare di cui sopra. Desidero pertanto chiederle, signor Ministro, quale sia l'indirizzo in termini di proposte e contributi, nonché lo stato di attuazione del pacchetto di iniziative a sostegno dei processi di economia circolare.

e dal progresso tecnologico, poiché occorre intervenire in tutte le fasi della vita del prodotto, le chiedo anzitutto cosa intende fare il Governo per promuovere, appunto, la ricerca nonché le *start-up* e le imprese a forte caratteristica innovativa in materia di riutilizzo e reimpiego di materia, con particolare riguardo alla utilizzabilità dei prodotti derivanti dall'agricoltura. chiedo se non ritenga opportuno incentivare gli enti locali a prevedere delle agevolazioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze, commerciali e non, che vogliono darsi gli strumenti per il ritiro dedicato di imballaggi non pericolosi. Ciò porterebbe ad una riduzione del quantitativo della della massa del rifiuto e contemporaneamente sarebbe da stimolo per il riuso.

se siete a conoscenza di tecnologie avanzate israeliane che prevedono l'eliminazione della raccolta differenziata, perché con la stessa tecnologia si è in grado di separare ogni tipo di rifiuto, anche l'umido.

vale anche per i prodotti agricoli a chilometro zero - c'è anzitutto bisogno di ingenti risorse, di cui non si vede adesso neanche l'ipotesi. È chiaro che è difficile,

cosa intende fare il Governo per poter sviluppare al massimo questa ipotesi che ci porta a emissioni zero rispetto alla produzione di energia, come da rapporto CETRI-TIRES. Questo è già documentato presso la Commissione europea ed è stato accettato dalla stessa. II Governo come si pone nel breve e naturalmente nel lungo termine (perché mi rendo perfettamente conto di ciò che serve)? Questa è la domanda cruciale rispetto al problema dell'economia circolare.

Signor Presidente, onorevoli senatori, è veramente importante il dibattito che stiamo svolgendo oggi sull'economia circolare e vi ringrazio per aver messo il tema al centro del *question time* odierno. Prendendo spunto dall'ultimo intervento svolto dal senatore Tarquinio, credo che noi riusciremo ad avere un'economia circolare solo ed esclusivamente attraverso un cambio culturale.

ossia sostituire l'economia lineare del Novecento con l'economia circolare del ventunesimo secolo. Ci vorrà tempo perché ciò implica un cambio molto profondo, che va dal singolo cittadino al grande imprenditore. Ognuno si deve sentire appartenente a questo processo che, come tutti i processi di grande trasformazione, ha bisogno di un cambio culturale e di un vantaggio economico. fa il senatore Di Biagio lo ha detto bene, ricordando le grandi tappe che sono state fatte nel 2015, che spingono tutte verso questo obiettivo. Occorrono, quindi, cambio culturale, da una parte, e vantaggio economico, dall'altra.

agevolare il percorso verso l'economia circolare, però ritengo che, oggi come oggi, abbiamo intrapreso una strada irreversibile. Tocca a noi stabilire la velocità con la quale vogliamo percorrere questa strada. Dobbiamo essere anche realisti, perché - ripeto - il percorso è di cambiamento radicale e credo che determinati passi richiedano tempo.

direttiva europea, la quale vedrà la luce probabilmente fra qualche mese. Abbiamo inteso anticipare i tempi proprio perché riteniamo che

con il Senato per giungere ad una chiara posizione italiana sul pacchetto dell'economia circolare, che sia condivisa non solo dal Governo ma anche dal Parlamento, in quanto ritengo che ciò sia di grandissima importanza.

e, in continuità con il percorso allora sviluppato, partecipa in maniera convinta ed intensa al dibattito sul tema a livello sia nazionale, che sovranazionale. Mi preme evidenziare come sia stato istituito un gruppo interdirezionale a carattere informale proprio all'interno del mio Ministero che esplica la sua attività specificatamente sul tema dell'economia circolare e dell'uso efficiente delle risorse. I due temi sono strettamente collegati. Già da settembre, in occasione della consultazione bilaterale con la Commissione europea, è stato istituito anche un tavolo tecnico di confronto con le altre amministrazioni coinvolte ed in particolare con il Ministero dello sviluppo economico. Tra le azioni che il mio Ministero sta portando avanti per favorire il percorso verso un'economia di tipo circolare, devono essere menzionate quelle volte all'attuazione di due importanti previsioni

per gli acquisti pubblici della pubblica amministrazione, e poi del GPP, il *green public procurement* che è una parte molto importante della partecipazione del pubblico all'economia circolare. Tramite questo strumento, le pubbliche amministrazioni sono portate ad integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto al fine di incentivare la diffusione di tecnologie e lo sviluppo di prodotti particolarmente pregevoli dal punto di vista ambientale. I CAM, cioè i criteri ambientali minimi, la cui adozione è diventata obbligatoria proprio ai sensi dell'articolo 18 del collegato ambientale, nonché ripresa nel testo di decreto legislativo di recepimento della direttiva appalti approvata proprio questa mattina in Consiglio dei ministri, prevedono infatti, per diversi tipologie di prodotti e servizi - carta per copie, cartucce per stampanti, arredi per ufficio, servizio di gestione dei rifiuti urbani, servizio di giardini, arredo urbano, tessili, ristorazione collettiva il possesso di specifiche caratteristiche tecniche in grado di favorire il recupero di materie di riuso. Proprio stamattina abbiamo approvato il decreto legislativo in materia di appalti in cui sono contenute grandissime novità in campo ambientale. C'è un processo di semplificazione per le bonifiche e una partecipazione del Ministero dell'ambiente attraverso il concerto sulle linee guida per la progettazione di tutte le opere pubbliche, quindi non più solo per le opere pubbliche che riguardano l'ambiente - bonifiche, depurazione acqua e rifiuti - ma anche quando si tratta di edifici e strade. Per la prima volta c'è il concerto del Ministero dell'ambiente sulle linee guida sulla progettazione, cosa che prima non esisteva, il che vuol dire che l'ambiente entra a pieno titolo anche nel capitolo delle grandi opere pubbliche. C'è poi una terza questione che riguarda l'economia circolare, cioè l'estensione a tutte le gare di appalto dei cosiddetti criteri ambientali minimi e quindi della soddisfazione di una percentuale di prodotti che tutte le amministrazioni (non solo Stato, Regioni e Comuni, ma tutte quelle che rientrano nel perimetro statale) devono tenere in considerazione quando fanno i propri appalti. Sempre nell'ambito delle recenti indicazioni contenute nel collegato ambientale, vanno pure ricordate le attività che il mio Ministero, attraverso il gruppo di lavoro interdisciplinare, porterà avanti in vista dell'attuazione degli articoli 21 e 23 di tale atto normativo. Queste attività, che vedranno anche il concerto degli altri Ministeri, riguarderanno principalmente l'approvazione di un piano d'azione nazionale

la Commissione europea ha presentato il nuovo pacchetto europeo sull'economia circolare in cui si analizza l'interdipendenza di tutti i processi della catena del valore, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, alla produzione, alla distribuzione, dal consumo al riuso e al riciclo. Contestualmente all'adozione del pacchetto pacchetto elaborato dalla Commissione europea contenente il piano per l'economia circolare sono state presentate quattro proposte di modifica delle direttive che ricadono nell'ambito del pacchetto delle misure dell'economia circolare. Le direttive oggetto di modifica sono quella che riguarda la discarica dei rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, i veicoli fuori uso e un'altra relativa alle pile, agli accumulatori e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nella giornata di domani i Ministeri dell'ambiente europei - proprio alla fine del *question time* partirò per Bruxelles - saranno chiamati ad esprimersi sul tema dell'economia circolare. Al riguardo si segnala che le proposte di modifica concernenti il pacchetto rifiuti non saranno oggetto di discussione nella sede del Consiglio, il quale sarà chiamato, invece, ad esprimersi unicamente sulle azioni previste dal piano sull'economia circolare. Sulla base degli esiti, dei dibattiti consiliari e delle discussioni in sede di Gruppo ambiente verranno elaborate e presentate al Consiglio ambiente di giugno le conclusioni del piano. In questa sede, in continuità con quanto già fatto, non mancheremo di segnalare importanti priorità, quali, ad esempio, la necessità di mettere in piedi azioni coerenti con lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde. prime seconde. Va evidenziato inoltre, che il buon esito di tale azioni dipende anche da una revisione della legislazione sui rifiuti, volta, tra l'altro, a rimuovere i principali ostacoli alla loro conversione in risorse. Sul punto è risaputo come una corretta applicazione della gerarchia delle fonti prevede innanzitutto attività di prevenzione.

in questo quadro si colloca il massiccio ricorso al conferimento in discarica che ancora si verifica in significative parti del territorio nazionale e a cui si dovrebbe ricorrere solo in via residuale.

Il Paese, nella raccolta differenziata, si presenta ancora a macchia di leopardo. Abbiamo zone in cui la raccolta differenziata ha raggiunto livelli europei e zone - lo voglio dire con estrema chiarezza - che sono da vergogna a livello europeo. Abbiamo ancora un conferimento in discarica troppo alto,

l'acronimo CAM, ovvero il criterio ambientale minimo, per definire le opere pubbliche, anche non ambientali, con criteri di qualità,

Da questo punto di vista mi dichiaro dunque soddisfatta e attendo di poter leggere e di conoscere le risposte puntuali, relative ai due quesiti che avevo posto, relativi all'*end of waste*, con i criteri che si chiedono di applicare immediatamente alle imprese italiane, e alla necessità di mettere a punto una legge quadro sui rifiuti.

Italia (impianti imposti come strategici), mentre è permissivo con la prevenzione e il recupero e fissa il tetto massimo di raccolta differenziata al 65 per cento, che per legge è invece un obiettivo minimo. Si tratta di una scelta politica che che risponde alle *lobby* degli inceneritori, che sono incentivati in un sistema di concorrenza sleale rispetto alle altre filiere. [DI

per la definizione delle misure in tema di promozione dei processi di economia circolare è stato molto proficuo. Mi sembra che il Governo abbia ben compreso l'importanza di questa sfida globale sulla quale il Ministero sta investendo molto come obiettivo successivo alla grande Conferenza COP21 di Parigi,

ringrazio il Ministro perché dalla sua relazione si evince l'impegno che il Governo italiano e il suo Ministero stanno profondendo affinché si realizzi l'economia circolare in cui ritengo che tutti ormai crediamo.

Naturalmente le difficoltà saranno principalmente di natura finanziaria, perché abbiamo il problema delle discariche, le risorse sono scarse e le discariche vanno quanto più possibile eliminate.

una parte importante dei rifiuti elettrici ed elettronici generati in Italia finisce ad operatori che, seppure in possesso dell'autorizzazione al trattamento dei RAEE (oltre 700 quelle rilasciate), si concentrano sulle materie prime seconde più semplici da estrarre e più remunerative. La situazione descritta ha come conseguenza la perdita per il sistema industriale di tutte le materie contenute nei RAEE, che vengono gestite in modo non corretto, e la difficoltà ad operare dell'industria virtuosa del riciclo dei RAEE che rispetti gli standard di trattamento esistenti. A tale difficoltà va aggiunto il recente crollo dei prezzi di mercato delle materie prime, stimabili nel 30-35 per cento da maggio ad oggi, rendendo vani gli appelli all'avvio dell'economia circolare. In questo quadro, uno dei passaggi necessari per dare slancio al settore della gestione ecocompatibile dei RAEE sarebbe l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 49 del 2014, secondo il quale «il Ministro dell'ambiente (...) determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento...». Tale decreto attuativo garantirebbe un livello omogeneo di qualità nel trattamento dei RAEE e controlli adeguati, consentendo a tutti gli impianti di trattamento di operare sulla base dei medesimi standard qualitativi. Rispondendo questa mattina a un'interrogazione presentata da me e da altri ventiquattro senatori, il Ministero ha affermato di non essere in grado di emanare questo decreto, perché la Commissione europea non ha ancora espletato alcune procedure preliminari. Ciò premesso, chiedo che se, nelle more dell'adempimento comunitario, il Ministero non possa in realtà promuovere con estrema urgenza iniziative, anche di tipo normativo, necessarie affinché la sostanza degli adempimenti richiesti nel suddetto decreto trovi immediata ed effettiva attuazione, anche in considerazione del fatto che le norme minime di trattamento per le differenti tipologie di RAEE sono già state pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. Credo che l'Europa abbia bisogno di una spinta anche dall'Italia, come sottolinea spesso il nostro Presidente del Consiglio. Signor Presidente, il fenomeno della bonifica dei siti produttivi è conseguente alla crisi profonda del nostro sistema industriale, che precede persino il recente tracollo economico-finanziario. Il lungo elenco di oltre cinquanta siti di interesse nazionale

Porto Marghera, Massa e Carrara, il Litorale Domizio e l'Agro Flegreo, Frosinone, gli interventi sui fiumi Saline ed Alento, ora nelle responsabilità della sola Regione Abruzzo (e non si capisce perché). Questi sono solo alcuni esempi di come la gestione delle bonifiche lascia spesso l'impressione di una totale irrazionalità.

attuale e preoccupante. Da recenti audizioni in Parlamento abbiamo capito come la responsabilità delle bonifiche sia spesso aliena da rigide logiche imprenditoriali. Abbiamo visto quantificazioni dei costi per gli interventi di bonifica assolutamente disancorate dalla realtà ed enormi sono le risorse sinora impegnate per le bonifiche dei siti di interesse nazionale. Signor Ministro, le chiedo dunque: qual è il criterio con cui si valutano le risorse pubbliche da destinare alla bonifica? Viene valutato un *business plan* iniziale? Esistono linee guida generali e comuni? Vengono posti precisi precisi doveri nell'affido dell'opera di bonifica? Esiste un controllo rigoroso delle risorse pubbliche impiegate e una verifica sui risultati?

Signor Presidente, signor Ministro, che il territorio italiano rappresenti il principale punto di approdo dei migranti, insieme alla Grecia, è un dato di fatto, come i problemi che inevitabilmente questo flusso crea. Uno di essi è proprio lo smaltimento dei barconi dei migranti utilizzati per la traversata. Da una mia recente ispezione al porto di Pozzallo ho potuto constatare come il Governo consideri queste barche dei rifiuti speciali, privilegiando la distruzione e lo smaltimento a carico dello Stato piuttosto che l'effettivo percorso di recupero, spesso possibile ed auspicabile. Ci risulta infatti che la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri datata 13 febbraio 2003 e rubricata «Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina», prevede la possibilità di procedere, in mancanza di istanze di affidamento avanzate dagli organi di polizia o da altri organi dello Stato, alla distruzione dei mezzi sequestrati. Considerato che lei, in occasione dell'audizione svolta presso il Comitato Schengen, ha dichiarato che non sarebbe scorretto parlare di dare vita a una filiera produttiva che possa garantire il recupero dei barconi stessi, potrebbe illustrarci quali misure il Governo sta adottando o intende adottare per rendere concreto questo progetto che appunto consisterebbe nel recupero delle stesse imbarcazioni e nel recupero dei materiali riciclabili e riusabili di quelle barche?

Signor Ministro, le sottopongo due questioni. Nella giornata di mercoledì 24 febbraio, i vertici aziendali di Caffaro Brescia Srl hanno annunciato ufficialmente che nel marzo 2017 lasceranno definitivamente il sito industriale di via Milano. Si apre, quindi, un problema occupazionale per le 55 persone che ancora ci lavorano, ma soprattutto un problema di sicurezza della falda acquifera legato allo storico inquinamento di policlorobifenile, prodotto dalla vecchia proprietà. L'attuale proprietà, come da accordi presi, ha l'obbligo di pompare e filtrare oltre un miliardo di litri di acqua dalla falda più profonda, per impedire che questa vada a contatto con quella più superficiale, totalmente inquinata dai veleni introdotti dalla Caffaro nel corso degli anni. Il proprietario aveva chiesto delle agevolazioni alle tariffe elettriche che doveva pagare, pari a un milione di euro l'anno. Gli sconti del Ministero non sono mai stati concessi. Al contrario, gli è stato chiesto di perfezionare il sistema di controllo, che fa acqua da tutte le parti, tanto che una relazione dell'ARPA ha certificato che ancora oggi l'inquinamento dei terreni a sud del sito Caffaro prosegue con lo sversamento di oltre 478 chili all'anno di veleni. Cosa succederà ora? Chi pagherà questi costi? Quale sicurezza per la salute dei cittadini? Italia dei Valori sollecita il Governo affinché adotti da subito provvedimenti di messa in sicurezza e poi provveda alla definitiva bonifica della Caffaro, stanziando le risorse più volte promesse dal suo Ministero ma ancora oggi non arrivate a destinazione. Altra questione riguarda l'ILVA. Lei sa benissimo che l'ILVA si salva solo a condizione di realizzare le bonifiche previste. Invocare la chiusura dell'ILVA ci sembra pura follia. Italia dei Valori ritiene che esista una strada percorribile: una *newco* che veda la Cassa depositi e prestiti al centro delle alleanze, anche internazionali, per realizzare un piano industriale composto dalle bonifiche, dalla innovazione del prodotto e dai nuovi impianti. Tutto questo vale circa tre miliardi, ed è l'unico criterio che per noi tiene insieme gli interessi del sistema industriale italiano con la sacrosanta difesa della salute delle persone che vivono a Taranto, unitamente ai posti di lavoro. Le chiediamo,

*(AP (NCD-UDC))*. Signor Ministro, la questione attinente alla virtuosa gestione dei rifiuti, con la conseguente gestione delle bonifiche dei siti di smaltimento degli stessi, riveste senza ombra di dubbio una rilevanza fondamentale per il nostro Paese. Molti, troppi, sono stati gli abusi e le violenze commessi ai danni del territorio e dell'ambiente, lasciando ancora oggi ferite aperte che dobbiamo rimarginare. L'atteggiamento era quello di voltarsi dall'altro lato e, utilizzando una metafora quanto mai calzante, di nascondere la polvere sotto il tappeto. Oggi, fortunatamente, si è arrivati ad una inversione di tendenza. Si è capito, in un'ottica più sensibile ai problemi ambientali, che il rifiuto può essere una vera e propria risorsa. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere visto come una opportunità di sviluppo, attraverso il recupero dei materiali, il loro riciclo e riuso, e la loro trasformazione in energia. Devo dare atto, signor Ministro, che da parte del suo Dicastero vi è stato e vi è un impegno forte

Un lavoro reso più difficoltoso, in molti casi, dalle lentezze burocratiche, dalla mancata partecipazione di alcune Regioni alle conferenze dei servizi, e perfino dai ritardi nell'emissione di quei provvedimenti preliminari e necessari, da parte delle Regioni, che consentono poi al Ministero di emettere i decreti di approvazione dei progetti di bonifica. Desidero pertanto chiederle, signor Ministro, lo stato dell'arte del lavoro compiuto sul fronte delle bonifiche relativamente ai progetti di bonifica approvati e ai decreti di autorizzazione di avvio lavori emessi. Signor Ministro, come è noto, dal 2001 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste e dal 2013 l'area industriale di Trieste è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali, nonché del recupero ambientale. Relativamente ai lavori di riconversione industriale della Ferriera di Servola, ricompresa nell'area appena descritta, in precedenti atti di sindacato ispettivo da me presentati ho chiesto delucidazioni circa la realizzazione di un nuovo laminatoio all'interno dello stabilimento, in particolare riguardo alle procedure autorizzative di inizio lavori in considerazione della peculiare situazione ambientale che caratterizza il sito in oggetto. Come si evince dal verbale della Conferenza dei servizi istruttoria, convocata presso il Ministero dell'ambiente in data 5 ottobre 2015, l'ARPA chiedeva un protocollo operativo in accordo con la Provincia competente per la verifica dei flussi sulla movimentazione dei materiali, ma soprattutto chiariva che non dovevano essere effettuate movimentazioni suolo e sottosuolo prima dell'emanazione del decreto di approvazione. Tali movimentazioni, invece, sono avvenute e sono dimostrabili come specificato da una mia precedente interrogazione. Considerato che il 2 novembre 2015 il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello stabilito che «nelle aree interessate dei rifiuti interrati, le opere previste devono essere avviate solo dopo la verifica dell'avvenuta completa rimozione dei rifiuti medesimi da parte degli enti locali di controllo» e che «deve essere concordato un protocollo operativo con la Provincia competente con la Provincia competente e l'ARPA per la verifica dei flussi sulla movimentazione dei materiali rispetto alla realizzazione del capannone o qualsiasi altra movimentazione all'interno dello stabilimento», le chiedo, signor Ministro, visto quanto esposto, se siano state disposte le opportune verifiche ispettive al fine di accertare la corretta esecuzione di inizio lavori del laminatoio in fase di costruzione nel rispetto del decreto ministeriale citato, nonché i risultati di eventuali esplorazioni di rifiuti interrati

nazionale (SIN) di Gela è stato istituito con la legge n. 426 del dicembre 1998. Il piano di disinquinamento per il risanamento ambientale prevedeva un totale di 47 interventi, di cui 14 a carico delle aziende e 33 a carico dello Stato. Nel 2000 il piano è stato commissariato, ma 17 anni dopo l'istituzione del SIN il territorio è ancora ben lontano dall'essere bonificato. Oltre agli enormi ritardi nell'esecuzione del risanamento, si è manifestata un'*escalation* preoccupante di patologie anche neoplastiche. Ad aggravare la situazione si sono aggiunti i problemi lavorativi degli operai legati all'indotto. I dipendenti delle imprese appaltatrici sono infatti fermi da tre anni e chiedono l'avvio dei cantieri per la riconversione *green* della raffineria, passando dal petrolio alla produzione di biocarburanti. Sappiamo che ci sono stati molti incontri, i quali finora hanno prodotto solo una proroga limitata della cassa integrazione. Si chiede, pertanto, signor Ministro, di conoscere lo stato dell'arte della bonifica riguardante il sito di Gela e se non ritenga utile attivarsi affinché il Governo trovi una soluzione definitiva per i lavoratori interessati, prevedendo, per esempio, una formazione dedicata, per riconvertire la loro professionalità in competenze da impiegare nelle concrete attività di bonifica.

Signor Presidente, proverò sommariamente a dare una risposta, perché i temi che avete sollevato sono tanti ed ognuno di essi richiederebbe un approfondimento

e i siti di gestione e smaltimento dei rifiuti. Il Ministero dell'ambiente è l'amministrazione competente per la predisposizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel perimetro dei quaranta siti di interesse nazionale. La legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha previsto l'istituzione di un Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento degli interventi e il trasferimento delle risorse. In attuazione della citata legge il mio Ministero, con decreto del 18 settembre 2001, ha adottato il regolamento recante il Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ripartire tra i siti di bonifica di interesse nazionale all'epoca già individuati le risorse disponibili.

In aggiunta a tali risorse, il Ministero ha assegnato a favore dei SIN ulteriori finanziamenti, a valere su risorse ordinarie di bilancio, risorse del Fondo di sviluppo e coesione (ex FAS) attribuite proprio al Dicastero dell'ambiente, risorse derivanti da atti transattivi stipulati con soggetti economici operanti sui siti inquinati. Quindi c'è una somma di risorse proveniente da vari capitoli. Le risorse complessivamente stanziate dal mio Ministero per interventi di bonifica di competenza pubblica nei SIN ammontano ad oggi a circa 2 miliardi di euro, che sono già stati trasferiti alle Regioni, ai commissari delegati e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ricordo che c'è un impegno da parte del Governo anche per gli ex SIN, per oltre 152 milioni, già trasferiti ai soggetti beneficiari. Quindi in totale sono 2.152 milioni di euro, molti dei quali sono già stati spesi, mentre altri sono in via di realizzazione degli interventi. Più in generale, le risorse sopra richiamate sono state disciplinate attraverso il ricorso a strumenti di programmazione negoziata, Accordi di programma e Accordi di programma quadro, sottoscritti dal Ministero con le Regioni, gli enti locali e le amministrazioni centrali coinvolte a vario titolo nel procedimento di bonifica, ovvero mediante l'emanazione di di appositi atti di disciplina a livello regionale o secondo le modalità previste nelle diverse ordinanze di Protezione civile nelle aree interessate. Il monitoraggio sull'attuazione del citato Programma nazionale è svolto, anche ai fini dell'attivazione della procedura di revoca dei finanziamenti, dalle Regioni, che provvedono annualmente a trasmettere al Ministero una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. Il Ministero, nell'ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario e di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore o ostativi la realizzazione dell'intervento, può proporre alla Regione competente l'adozione delle procedure di revoca o riassegnazione delle risorse. Sul SIN di Trieste ho tutta la storia scritta, ma mi limiterei, per brevità, a leggere la risposta diretta all'interrogante, relazione un po' tutta la storia del SIN, fino ad oggi. Sul quesito relativo al SIN di Trieste e sulle verifiche ispettive per l'esecuzione di inizio lavori del laminato nel rispetto del decreto di approvazione, si rappresenta che il controllo e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite con il decreto di approvazione degli interventi di cui al progetto integrato è di competenza degli enti di controllo locali, ai quali è attribuito il compito di verificare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'attuazione degli interventi. Tuttavia, alla data di avvio dei lavori propedeutici alla costruzione del capannone dove verrà allocato il laminatoio, il Comune di Trieste, successivamente alla Conferenza dei servizi del 5 ottobre 2015, che riteneva approvabile il progetto in questione, comunicava che i lavori relativi alla realizzazione del capannone industriale erano già stati avviati con l'esecuzione delle opere fondazionarie, dei pilastri e della relativa copertura. Pertanto la mia direzione, il giorno seguente, informava la Provincia di Trieste e l'ARPA competente al fine di accertare eventuali infrazioni alla normativa ambientale per le opere avviate. La Provincia, a riscontro della richiesta, comunicava la propria riserva nel valutare assieme ad ARPA quanto lamentato. Si segnala, infine, che con la nomina del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia quale commissario straordinario, avvenuta il 7 agosto 2015, è posta in capo allo stesso la responsabilità del monitoraggio e dell'attuazione degli interventi, sia per la parte privata che per Per quanto riguarda il SIN di Gela, do conto di tutta la impermeabilizzazione fatta, delle risorse che abbiamo stanziato e della storia complessiva del SIN, di cui rimanderei la lettura perché è molto tecnica e molto articolata, mentre mi sta a cuore parlare soprattutto delle procedure di infrazione in materia di discariche, questione sottoposta dal senatore Di Biagio e da altri interventi. In relazione al caso relativo alla mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva rifiuti, tenuto conto dell'intensa attività svolta dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con con tutte le altre amministrazioni coinvolte, si è passati da 200 discariche abusive, quelle oggetto della infrazione (che è del 2007, quindi si fa riferimento alla situazione in quel momento,

di 14 discariche ed un errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale. In data 8 febbraio 2016 la Commissione ha riconosciuto altresì la messa a norma di 29 discariche e un ulteriore errore di censimento, escludendo anche questi siti dal computo della penalità. Si fa presente, inoltre, che delle 155 discariche ancora oggetto di procedura, 151 sono state destinatarie di diffida da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio su impulso del mio Ministero, ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo, e per gli altri 4 sono in corso approfondimenti istruttori. Si ricorda, peraltro, che il Ministero dell'ambiente ha adottato uno specifico Piano straordinario di bonifica relativo a 45 discariche, in attuazione proprio dell'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2014. Al riguardo, è stata assegnata la massima priorità agli interventi in aree di discariche pubbliche ritenute cantierabili nelle Regioni interessate. Con le risorse disponibili per l'attuazione del citato piano sono stati immediatamente finanziati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica relativi a 26 discariche ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Puglia, Sicilia e Veneto, disciplinati in specifici Accordi di programma, prevedendo che l'erogazione delle risorse assegnate avvenga subordinatamente alla presentazione dei quadri economici definitivi degli interventi. Al riguardo si segnala che ad oggi non è pervenuta alla competente direzione generale la predetta documentazione, pertanto non risultano ancora trasferite le risorse. Le restanti 14 discariche, allo stato, sono inserite nella fase programmatica del suddetto Piano straordinario. I relativi interventi potranno, pertanto, essere attivati non appena reperite tutte le risorse necessarie. Ad ogni modo, si ricorda che con la legge di stabilità 2016 è stato finanziato, per un importo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, il fondo di cui al citato articolo 1, comma 113. Per le 155 discariche in procedura di infrazione è stato stimato un fabbisogno finanziario complessivo, sulla base dei progetti disponibili presso i Comuni e le Regioni competenti, pari a circa 290 milioni di euro per i relativi interventi tecnici programmati. Cosa abbiamo fatto noi? Rispetto allo stato dei procedimenti in corso, per le 155 discariche ancora oggetto della procedura di infrazione, come già evidenziato, segnalo che sono state notificate alle Regioni e agli enti locali interessati 151 decreti di diffida, che per quattro sono in corso approfondimenti istruttori. Per ogni singolo procedimento di diffida sono stati definiti termini congrui per l'espletamento delle attività e sono attualmente in corso le attività di monitoraggio delle stesse. Mi permetto di dire che su questo dato andrebbe fatta una riflessione, perché questo non è il modo normale di operare: 151 diffide vuol dire che c'è qualcosa di strutturale che non funziona, perché il mio Ministero non è fatto per surrogare gli enti locali o le Regioni, ma per esercitare un potere di controllo e di indirizzo. Allora, se io mi trovo nel campo dei rifiuti, delle bonifiche, della depurazione, a dover esercitare continuamente i poteri sostitutivi,

I termini imposti nelle diffide non sono tutti scaduti e la situazione è quotidianamente monitorata dal mio Ministero. In dieci casi gli enti territoriali hanno adempiuto a quanto richiesto nei termini imposti tutto ciò si raccoglie la documentazione, al fine della trasmissione alla Commissione europea per il calcolo della terza sanzione semestrale. Sarà impegno del mio Ministero proseguire nel cospicuo lavoro di impulso e monitoraggio delle diverse amministrazioni locali. Mi piace ricordare che il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di legge di stabilità, di una norma volta a rendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato, a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui

la legge di stabilità ha previsto una novità: è stato attivato un meccanismo di compensazione con i trasferimenti che lo Stato deve effettuare alle Regioni responsabili della violazione in base alle sanzioni, compensazioni per le quali non sarà più necessario acquisire l'intesa delle amministrazioni locali e regionali coinvolte. ed elettroniche (RAEE), sollevata dal senatore Dalla Zuanna, in particolare in merito all'attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, come ricordava lo stesso senatore, il sottosegretario Degani ha già avuto modo di riferire alle Commissioni ambiente. Farei pertanto a meno di ripetere la risposta di questa mattina, però sono pronto a prendere in seria considerazione l'impulso che viene dal senatore Dalla Zuanna e da tutti i senatori che hanno presentato che hanno presentato l'interrogazione per vedere in quale modo possiamo anticipare le decisioni dell'Europa perché il problema è reale, esiste. Bisogna vedere, dal punto di vista normativo, quali possibilità di intervento abbiamo a questo fine. Per quanto riguarda il problema della Caffaro-Brescia srl, sapete che c'è un'attenzione particolare del Governo su questo tema.

a valere sul decreto ministeriale n. 308. Le predette risorse sono già state tutte trasferite alla Regione Lombardia e

È stata quindi trasferita a favore della Regione Lombardia un'ulteriore somma di 1.106.064 euro. Successivamente all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi previsti nel sopracitato Accordo di programma,

euro, ho già ribadito più volte che tali risorse sono state chieste sulla programmazione delle risorse europee 2014-2020 e confido che possano arrivare in tempi brevi.

fondamentali per la vita di migliaia di famiglie. L'augurio, quindi, è che anche le bonifiche industriali, così come la gestione dei siti di smaltimento dei rifiuti, non diventino un affare troppo costoso per i contribuenti italiani, un'occasione troppo facile per le mafie ed un problema che, come troppo spesso accade in Italia, si trascina per anni perennemente irrisolto.

In particolare, ritengo che l'utilizzo dei barconi possa diventare uno strumento utile per aumentare le opportunità lavorative, non solo dei pescatori dei territori delle zone di prima accoglienza, ma di tutti quei privati disposti ad intraprendere attività di turismo nel proprio territorio. Tra l'altro, si potrebbero così evitare i costi di smaltimento in discarica che pesano sulle casse dello Stato. Qualcuno mi ha anche consigliato di pensare al recupero dei barconi per soddisfare finalità di decoro monumentale e museale, di cui potrà godere certamente tutto il territorio nazionale. Qualche cooperativa siciliana mi ha perfino suggerito di piazzare alcune di queste barche nei parchi giochi dei bambini, così da diventare strumenti ludici ed educativi che rafforzino la memoria delle tante stragi avvenute nel nostro territorio e nel nostro mare.

che il confronto di oggi possa essere utile al fine di attirare sempre di più l'attenzione su problematiche che hanno effetti diretti ed immediati sulla vita dei nostri cittadini. Sono soddisfatto di quanto lei oggi ci ha detto, dimostrando ancora una volta la grande determinazione di questo Governo a mettere in atto tutte le misure che possono condurre verso un miglioramento della qualità dell'ambiente.

comunque, c'è sempre una responsabilità di chi gestisce il territorio, delle Regioni, dei Comuni e di chi non fa effettivamente i controlli, oltre che la noncuranza e l'illegalità di chi è amministratore e proprietario delle aziende che hanno questo tipo di atteggiamenti.

Signor Presidente, ringrazio il Ministro della risposta. Parliamo di un sito dove ci sono state 3.000 tonnellate di rifiuti tombati e il tombamento è comunque l'ammissione di una sconfitta delle precedenti amministrazioni, com'è stata gestita l'attività industriale e soprattutto ambientale in quell'area. Al momento ci sono altrettante migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi ancora da smaltire. Ribadisco la mia preoccupazione sulle autorizzazioni che sono state accordate dagli enti preposti per la costruzione del nuovo capannone, perché dalla sua risposta si evince che i lavori sono avvenuti prima dell'emissione del decreto interministeriale, che data 2 novembre. Questo ci fa apprezzare quanto lei ha detto, perché ovviamente servirebbe un maggiore collaborazione ed un maggiore impegno degli enti locali per monitorare quello che avviene nel nostro territorio. Mi dispiace tuttavia

cui la prego di prestare attenzione, verificandone la fattibilità: da un lato abbiamo le bonifiche da fare sul sito di Gela e dall'altro abbiamo operatori che rischiano di essere licenziati per mancanza di lavoro.

fino a Trapani e parlare dei problemi locali è l'errore più grave che si possa fare. La problematica è complessiva e quindi va affrontata complessivamente, per insisto che sia affrontata a livello nazionale. La consapevolezza del Ministro mi rende fiducioso rispetto a ciò che sarà. Le risorse necessarie sono enormi, i soldi in Europa ci sono, qualche altra cosa potremo fare, ma credo che la strada giusta sia stata intrapresa. molta collaborazione l'attività del Ministro e poi, tutti quanti, giudicheremo.